L'ordine del giorno reca la discussione del relazione della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari sulla elezione contestata nella circoscrizione Estero del senatore Nicola Paolo Di Girolamo. La Giunta ha deliberato di proporre al Senato l'annullamento dell'elezione del senatore Di Girolamo. La relazione è stata stampata e distribuita. Chiedo ai relatori, senatori Augello e Li Gotti, se intendono intervenire per integrare la relazione scritta.

Presidente, onorevoli colleghi, siamo qui ad esaminare un caso complesso e delicato. Voglio in primo luogo dare atto alla Giunta delle elezioni di aver compiuto un esame Non possiamo però in questo momento così importante dimenticare che i fatti in ordine ai quali è stato aperto il giudizio di contestazione sono anche oggetto di un procedimento penale penale pendente nei confronti dello stesso senatore. L'esistenza delle indagini in corso ovviamente non incide sull'autonomia decisionale e l'indipendenza del giudizio del Senato. Ricordo infatti a questo proposito che l'Assemblea si è pronunciata - è un dato di grande rilievo per tutti noi - in data 24 settembre 2008 in senso contrario all'autorizzazione dell'esecuzione della misura cautelare degli arresti domiciliari avanzata dal giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Roma, un'iniziativa ancora pendente che in quanto tale comporta una decisione non solo sul tema specifico che la Giunta ha già approfondito, ma anche su una situazione rispetto alla quale il Senato si è espresso recentemente negando l'autorizzazione all'arresto. Tuttavia, devo anche richiamare l'attenzione dei colleghi sulla considerazione che, ai fini di una piena e serena valutazione della vicenda, è necessario tenere conto di tutti i complessi e delicati profili della questione, tra i quali rientrano anche gli sviluppi del giudizio penale sui fatti in oggetto. Pertanto, riteniamo che, tenuto conto della richiesta di arresto della decisione presa dal Senato il 24 settembre 2008 contro l'arresto, la decisione odierna abbia una sua ulteriore rilevanza. Perconsentire all'Aula un esame più approfondito dell'argomento all'ordine del giorno, anche alla luce di un'ulteriore valutazione che la magistratura potrà formulare nell'ambito delle proprie competenze,

Stiamo applicando l'articolo 66 della Costituzione che, a differenza di molti altri Parlamenti nel mondo, attribuisce alla nostra Camera il potere e il dovere di valutare i titoli di ammissione di ciascuno di noi all'esercizio della funzione parlamentare.

i giudici chiamati a decidere l'ultimo atto di un procedimento giurisdizionale assegnato esclusivamente alla nostra cura da parte della Costituzione; pertanto non possiamo

Colleghi, ho ascoltato la richiesta del presidente Gasparri e l'intervento del senatore Sanna. Ritengo che la questione sospensiva sia un istituto di carattere generale,

per le ragioni che espongo brevemente. L'unica fonte regolamentare della fase decisionale che siamo chiamati ad affrontare questa mattina

che almeno 20 senatori non presentino un ordine del giorno motivato in difformità della decisione della Giunta medesima. Questa è la norma regolamentare.

pregiudiziale è un istituto di carattere generale e che quindi si applicherebbe ad ogni sorta di deliberazione dell'Aula del Senato. A nostro modo di vedere, le cose non stanno così, per le ragioni che ha esposto il senatore Sanna, ma anche per ulteriori ragioni molto evidenti, riconducibili a due ordini di argomentazioni: la prima è che la norma di cui all'articolo 93 del Regolamento è dettata esclusivamente nell'ambito del procedimento legislativo la seconda è che, se così fosse, o meglio se la tesi sostenuta dal presidente Gasparri venisse da lei accolta, si configurerebbe una sorta di doppio grado di giudizio, nel senso che l'Aula del Senato sarebbe chiamata

che una questione identica a quella proposta dal presidente Gasparri (è questo è un dato molto rilevante, a mio modo di vedere) fu posta durante il procedimento davanti alla Giunta. La difesa del senatore Di Girolamo,

senso di respingere queste questioni e, anzi, la questione pregiudiziale penale, se mal non ricordo, fu ritirata dalla difesa del Di Girolamo.

noi non possiamo in alcun modo accogliere la sua decisione. La invitiamo a rivederla alla luce delle argomentazioni che mi sono permesso di svolgere e, nel caso, ad investire della questione la Giunta per il Regolamento. Si tratta di una decisione che potrebbe costituire un precedente molto pericoloso, perché è evidente che ove fosse accolta l'attività paragiurisdizionale svolta dalla Giunta per le elezioni verrebbe totalmente svuotata di significato.

della maggioranza volessero porre una questione che attiene alla non condivisione nel merito della decisione della Giunta, (che è l'unico strumento disponibile per noi senatori), dovrebbero far rifluire questa tesi

per noi disponibile e l'unico che lei può ammettere alla votazione di quest'Aula. *(Applausi Senatore Legnini, sto cercando di ascoltare, doverosamente e con la massima attenzione, tutti gli interventi, perché si tratta di un caso estremamente delicato. Riscontro, senatore Legnini, l'esistenza di due precedenti su un'ammissione di questione sospensiva su un incardinamento di un parere della Giunta, del 1993 a carico del senatore Bargi e un altro del 2002 per il senatore Malentacchi. In queste occasioni, ad inizio di seduta vennero presentate delle proposte di sospensiva, che vennero votate. La invito poi ad esaminare

un richiamo alla sostanziale applicabilità, perché ove si fosse sostenuta una inibitoria della questione sospensiva qui vi sarebbe stato un richiamo *a contrario*.

Devo dire che il contesto, non solo regolamentare ma anche quello della prassi d'Aula, mi sembra univoco; non ho spunti né dal Regolamento, né dai precedenti per poter accedere ad una riflessione, pur con il massimo degli sforzi.

Presidente, stiamo affrontando una questione particolarmente delicata perché, al di là della vicenda concreta, alla quale ciascuno di noi ovviamente guarda con l'attenzione che merita, stiamo ragionando della possibilità - perdonatemi questo termine - di una interferenza in un procedimento, quello previsto dall'articolo 66 della Costituzione, da parte dell'Aula. Il riferimento che ella fa all'articolo 106 del nostro Regolamento,

Le osservazioni che il senatore Sanna faceva in apertura, ulteriormente corroborate non solo dalle osservazioni in punto di diritto fatte dal senatore Legnini, ma soprattutto da quelle in punto di fatto precisate dallo sono a mio avviso non sormontabili. Il senatore Legnini ha ricordato che la stessa richiesta che oggi il senatore Gasparri ha avanzato qui in Aula

particolare non trascurabile perché ovviamente toglie *vis* al passaggio d'Aula, che a questo punto vede la Giunta e la sua proposta come protagoniste dell'intero procedimento),

richiesta di sospensiva sono motivazioni che, fatte valere nel giudizio di Giunta, anche alla luce della precorsa decisione dell'Aula in ordine al respingimento della richiesta di autorizzazione a procedere all'arresto, avrebbero avuto un loro senso pieno; poste qui in Aula, non sono intralcianti: non potrebbero neanche essere formulate. Se la richiesta avanzata dal senatore Gasparri fosse stata consacrata in un ordine del giorno, presentato da almeno venti senatori, con un dispositivo difforme rispetto alle conclusioni della Giunta, saremmo nella piena vigenza del Regolamento e osserveremmo il rito speciale - diciamo così che viene attribuito al Senato in quanto giudice speciale e unico su tale materia. Ma fuori da questa forma, ritenere che qualunque strumento venga previsto dal Regolamento per regolare la discussione dei disegni di legge o di qualunque altro affare sia applicabile anche a questo giudizio secondo me è sbagliato. Il fatto che non abbiamo precedenti probabilmente illumina circa il fatto che ci troviamo davvero di fronte ad una richiesta eccentrica rispetto alla previsione e alla garanzia che nell'ordinamento I colleghi della maggioranza non possono assumere che in questo modo venga leso un diritto del senatore Di Girolamo, poiché lo strumento esiste ed è strumento speciale: l'ordine del giorno presentato da almeno venti senatori,

opinioni suffragate da impostazioni giuridiche diverse. Noi però, Presidente e colleghi, non siamo tanto interessati alle solite eccezioni, eccentriche definite da qualcuno, di ordine regolamentare. L'Italia dei Valori chiedere di conoscere se, a parere del Senato,

lo faccia, se ne assumerà la responsabilità, ma il mio Gruppo non è affatto interessato a discutere di queste cose in questo momento quando siamo già in Aula e dovremmo giudicare sulla sostanza, non su un formalismo vieto che probabilmente non interessa nessuno.

sua concretezza ed è stato posto da suoi colleghi dell'opposizione, oltre che da eminenti componenti della Giunta, e dunque è giusto che questo Senato lo esamini con la serietà che esso merita. merita. Sulla questione vi sono considerazioni che lei ha colto che ci portano a ritenere che essa non si ponga. In realtà, la generalità alla quale fa riferimento l'articolo 93 comprende Sarebbe, a nostro avviso, una *deminutio* per i poteri dell'Aula di serie conseguenze. Vorrei però aggiungere altri due elementi che fanno riferimento alle procedure che si sono svolte e non troppo tempo fa in questo Senato. prima riguarda, per l'appunto, la stessa Giunta delle elezioni, laddove, proprio su questo procedimento, in merito alla costituzionalità della norma che era in discussione, fu presentata una pregiudiziale. Non si tratta di una sospensiva ma, come sappiamo, da un punto di vista regolamentare fanno parte della stessa famiglia.

essa doveva essere riportata all'Aula ed era l'Aula il luogo nel quale essa avrebbe dovuto essere, eventualmente, presentata e discussa. Faccio poi riferimento ad un elemento che, secondo me, è ancora più stringente dal punto di vista anche dei nostri rapporti

io leggo che in merito all'elezione contestata nella circoscrizione estero, gli eventuali ordini del giorno in difformità, da presentare entro la fine della discussione generale, saranno votati a scrutinio segreto. Saranno invece poste ai voti per alzata di mano le semplice questioni sospensive. Queste decisioni sono state assunte all'unanimità, con tutti i presenti

anche per consentire ai Gruppi, nell'articolazione del loro dibattito interno, di tenerlo presente. Non è stato fatto. Queste sono state le regole del gioco fissate di comune accordo e questo, credo, è il gioco che oggi dobbiamo giocare. Non perché la questione posta sia un vieto formalismo, come crede il senatore Belisario, ma perché è stata considerata nella sua serietà, credo che potremmo arrivare al parere condiviso ed è giusto per tutti andare avanti con le regole che insieme abbiamo determinato. *(Applausi Trattandosi di un tema delicato, la Presidenza sarà ovviamente permissiva nella tolleranza nei confronti di tutti i colleghi.

precisò molto attentamente come il rapporto tra quella Giunta - tenete presente che noi, a differenza della Camera, abbiamo un'unica Giunta - e l'Aula doveva essere quello di non sovrapporre mai decisioni in sede di autorizzazioni a procedere con decisioni in sede di verifica dei poteri. Da questo punto di vista mi permetto di sottolineare l'opportunità della considerazione del senatore Gasparri. Quest'Aula nel settembre scorso si è pronunciata sulla vicenda in sede di autorizzazioni a procedere. Oggi ha all'ordine del giorno una questione di verifica dei poteri nella quale, qualora venisse accolta la proposta della Giunta, sovvertirebbe, a così breve distanza nell'arco di una stessa cronologia, una decisione presa dall'Aula. Il che, non voglio citare nessun precedente,

Grazie

e si pone il problema che in dottrina esistono opinioni diverse sulla limitazione dell'elettorato passivo, afferma che noi siamo in un procedimento del tutto speciale e siamo un giudice del tutto speciale. speciale. Non siamo un giudice qualsiasi che esamina posizioni dottrinali su questa materia: siamo il Parlamento della Repubblica che ha votato questa legge e che si è posto questi problemi quando ha votato la legge. Quindi, la specialità del procedimento è tutta in queste parole

articolo dice che è stato piegato da interpretazioni regolamentari e prassi politiche per autodifesa della classe politica e per rispettare la legge ferrea che chi entra in Parlamento non ne deve mai uscire, anche se non ne ha i titoli. Questo è quanto scritto non in saggi rivoluzionari o in arringhe di piazza, eppure questo è stato il modo con cui l'articolo 66 è stato piegato nella prassi. Se noi vogliamo delegittimare un pezzo di Costituzione con i nostri comportamenti

Presidente, non vorrei abusare della sua pazienza e di quella dei colleghi, ma forse vale la pena ribadire tre passaggi che non riusciamo a comprendere come non vengano portati adeguatamente all'attenzione dell'Assemblea. Il primo passaggio, Presidente, è contenuto nel resoconto della seduta pubblica della Giunta del 20 ottobre 2008, a pagina 16, dove espressamente, come già ricordato dalla mia Capogruppo e da altri colleghi intervenuti, il difensore del senatore Di Girolamo dice al Presidente di rinunciare alla pregiudiziale penale. Quindi, Presidente, la parte ha rinunciato espressamente, fino all'ultima seduta possibile, alla pregiudiziale che oggi è stata posta dal presidente Gasparri.

Il punto non è irrilevante perché la Giunta, dopo essersi espressa sulla questione di legittimità costituzionale in altro passaggio, avrebbe ben potuto esaminare la pregiudiziale penale in quella sede; non lo ha potuto fare, perché la parte interessata vi ha rinunciato. In secondo luogo, signor Presidente, Presidente, la Giunta, dopo un lavoro massacrante - mi si permetta di dirlo - che ha investito alcuni di noi per l'intero mese di agosto, è pervenuta ad una decisione sofferta e decisa, ma unanime, il 20 ottobre. oggi siamo alla fine di gennaio, sono passati tre mesi; è la prima volta che in Aula arriviamo per il perfezionamento di un procedimento, come previsto dal Regolamento del Senato;

non abbia chiesto in sede di Conferenza dei Capigruppo di parlare di questo tema dato che avevano intenzione di proporre la pregiudiziale penale. Perché far passare tre mesi, signor Presidente del Senato? Potevano farlo nei tre mesi precedenti e non lo hanno fatto.

il Capo XII, in un ordine logico e non opinabile - a meno che qualcuno non dimostri il contrario -, arrivi a trattare la fase di discussione di ciò che è in Aula. è in Aula. Tratta questa fase dopo che si è parlato dell'introduzione e dell'esame dei disegni di legge all'attenzione dell'Aula. Lei giustamente ha definito l'articolo 106 una norma di chiusura; ma, signor Presidente, mi permetto di ricordare a me stesso che questa norma di chiusura è, come lei ha detto, norma generale, ma le norme generali - dico sempre a me stesso - sono superate solo dalle norme speciali che derogano a quelle generali.

In questa fattispecie è l'articolo 135-*ter* a dovere essere applicato perché noi non siamo in un nuovo procedimento che duplica i lavori della Giunta, ma siamo in una fase di perfezionamento dei lavori della Giunta Stavo concludendo - la ringrazio ancora per la pazienza -, ricordando ciò che la presidente Finocchiaro ha detto pochi istanti fa. Signor Presidente del Senato, si poteva presentare un documento con 20 firme di senatori, che però non è stato presentato.

come è apparso inequivocabilmente davanti alla Giunta delle elezioni al Senato che, in data 20 ottobre, ha ordinato l'annullamento della sua elezione, rispettando così la nostra Costituzione. La lettera l'avete tutti

Grazie in virtù di un mandato popolare e che in questo momento sono dei giudici che devono verificare situazioni molto delicate e complesse. Domando a loro - a tutti e a ciascuno di loro - quanti hanno preso visione e sono consapevoli di tutti gli elementi precisi, di dettaglio, problematici, risolti o meno dalla Giunta delle elezioni, contenuti il punto è questo: noi oggi siamo chiamati a pronunciare una sentenza definitiva sulla base di elementi che, in tutta coscienza, dobbiamo verificare direttamente e personalmente. GARAVAGLIA Mariapia Per questo credo che una sospensiva, dettata da ragioni di opportunità (nel senso di una verifica del contenuto dei dati e degli elementi della relazione della Giunta), sia più che necessaria.

ho impiegato parecchie ore per leggere con attenzione la relazione e per analizzare tutti i punti in essa contenuti. Credo che la prima consapevolezza che dobbiamo assumere è che in questo momento, forse per la prima volta nella storia di questa Camera,

si debbano chiedere un approfondimento e una riflessione dei temi posti dalla Giunta delle elezioni. Presidente, non entro nel merito delle questioni regolamentari che sono state affrontate dal senatore Sanna, dal senatore Legnini e poi dalla presidente Finocchiaro,

dopo un'istruttoria che ha tenuto impegnati gli uffici, alcuni componenti della Giunta e i relatori in prima battuta per molte settimane e che si è conclusa nel mese di ottobre. Poiché l'argomento era all'attenzione di tutti e non soltanto dei membri della Giunta, io ricordo che quando si è trattato di decidere, avendo presente che c'è una lunga prassi parlamentare che induce a considerare con molta attenzione le ragioni dei colleghi che fanno parte dell'Assemblea e sapendo bene che sull'altro piatto della bilancia c'era il valore della legalità, la Giunta si è espressa all'unanimità senza sorta di distinzioni politiche, tant'è che i due relatori sono

Se in presenza di una decisione della Giunta adottata in punto di diritto e senza controversia politica e se a tre mesi di distanza viene introdotta comprensibilmente una tecnica dilatoria, che però frena una decisione che è stata condivisa da tutti i Gruppi politici, mi domando e domando al Parlamento se questa sia una pagina della vita parlamentare che induce a considerare con favore e a sottolineare la possibilità di intese *bipartisan*, come si usa dire, o se viceversa noi non stiamo mettendo un granello in più nell'ingranaggio già tanto farraginoso delle intese che con fatica i Gruppi realizzano nel lavoro parlamentare. Questa è la domanda che mi sento di fare e questa è la ragione per cui chiedo al Parlamento di decidere oggi in un senso o nell'altro avendo rispetto non soltanto del lavoro fatto dalla Giunta, ma dello spirito assolutamente equanime con cui tutti i componenti della Giunta, almeno quelli che sono stati presenti e che hanno votato allo stesso modo, hanno lavorato. *(Applausi dai

Presidente, l'intervento del presidente Follini mi induce a fare all'Aula una considerazione. Non stiamo mettendo in discussione soltanto le conclusioni unanimi della Giunta, come adesso ci ha ricordato il senatore Follini; noi stiamo mettendo in discussione il prestigio della Giunta. Stiamo mettendo in discussione il valore istituzionale delle decisioni della Giunta. Io vorrei richiamare l'Aula e lo dico, se mi permette l'espressione, con amicizia anche al presidente Gasparri: non metteteci nella condizione di dover chiedere da domani al Paese e al Parlamento di rivedere profondamente gli istituti che la nostra Costituzione ha posto a tutela dei parlamentari e del Parlamento; non metteteci in questa condizione. Non vogliamo chiederlo, ma ci state spingendo a farlo

davanti anche al tempo passato noi ci facciamo prendere dall'interesse politico e di parte per negare efficacia alle decisioni della Giunta delle elezioni, credo, signor Presidente, che a noi - e forse non soltanto a noi - dopo non rimanga che una sola possibilità: chiedere che venga levato al Parlamento il potere di assumere queste decisioni.

a seguito della decisione della Giunta, che noi non intendiamo mettere in discussione con questa richiesta di sospensiva, 80 senatori della Repubblica di questo Gruppo hanno sottoscritto un appello ai propri Capigruppo

che forse era il caso di assumere un elemento di riflessione. Signor Presidente, il senatore Compagna ha citato il caso del senatore Bargi. voglio ricordare a quest'Aula che, seppure colpito da una violenta ondata di fango, egli fu assolto da tutti i reati. Vorrei pure ricordare a quest'Aula un'esperienza personale che mi ha spinto dinnanzi ai miei figli qualche mese fa quasi a vergognarmi di essere

Vorrei che quest'Aula desse il tempo anche al senatore Di Girolamo di dimostrare la sua estraneità ai fatti che gli vengono contestati perché questo Paese è percorso

Signor Presidente, le assicuro che questo è un intervento che non avrei voluto fare.

e non dire ciò che sento, in quanto eletto nella circoscrizione Estero. La circoscrizione Estero non è un terreno selvaggio da conquistare. Gli italiani all'estero non sono persone da colonizzare e da utilizzare; non sono uno strumento. Gli italiani all'estero sono un pezzo dell'Italia ed hanno contribuito, insieme a tutti gli altri italiani, insieme a voi che siete rimasti in Patria, a fare l'Italia di oggi. Abbiamo contribuito lavorando lontano dall'Italia, ma lavorando per l'Italia. Qualsiasi strumento ampli i poteri in funzione della democrazia è importante. L'esercizio del voto all'estero e la presenza di parlamentari che provengono dalla circoscrizione Estero sono sicuramente un progresso della democrazia. Ma nella democrazia si può anche abusare. Ed è anche giusto poterlo fare, collega De Gregorio, perché lei ha creato un partito che si chiama «Italiani nel Mondo».

IdV).* Essere emigrante è altra cosa, senatore De Gregorio. Lei usurpa questo nome per farsi una clientela politica. Però, lei sa che non si può presentare all'estero!

a rimettere in questione il lavoro svolto dalla nostra Giunta. Oggi non dovevamo neanche dibattere o discutere. Se non c'è quell'ordine del giorno con venti firme non vuol dire qualcosa? Non vuol forse dire che non ci sono venti senatori che vogliono mettere la loro firma e il loro nome, la loro faccia in questa storia?

abbiamo fatto discorsi sugli stupri, sul rispetto delle leggi, sulla violenza negli stadi. Questo che viviamo oggi è uno stupro all'Aula, e io non vi partecipo. Colleghi, la Presidenza ritiene di avere le idee sufficientemente chiare sulla ammissibilità o meno della richiesta di sospensiva. Però, intendendo seguire tutti gli sforzi possibili ed immaginabili perché vengano

Grazie riprendiamo i nostri lavori. Alla luce dell'interpretazione regolamentare e dei precedenti, che sono tutti coincidenti e, tra l'altro, distanti più di dieci anni uno dall'altro (questo a confermare l'uniformità di una giurisprudenza interna),

Rimaniamo fortemente sconcertati per quella che riteniamo una forzatura del Regolamento in presenza di una sostanza definita all'unanimità che ha chiarito tutti i passaggi. Riteniamo una mortificazione per il Parlamento nascondere dietro

Poi ci lamentiamo della distanza tra Paese reale, intendendo i cittadini, e Paese legale, intendendo il Palazzo. Ma quando il Palazzo decide cercando di rimanere nella legalità (così ha fatto la Giunta delle elezioni arriva qualcuno che alla fine propone di sospendere, di fatto *sine die*,

delusa, rammaricata perché ritiene che il Paese non meriti i ceffoni

Presidente, abbiamo illustrato poc'anzi, attraverso gli interventi dei colleghi Sanna, Ceccanti, mio, dei senatori Lusi e Legnini, le ragioni per le quali noi crediamo che la sospensiva non possa essere accolta; anzi, *rectius*, che la sospensiva non possa essere posta in questa fase del procedimento. Vorrei però tornare su alcune questioni che certamente orienteranno la decisione dell'Aula. Mi pare fuori di dubbio che l'unico giudice, il giudice esclusivo di questa materia a norma dell'articolo 66 della Costituzione, la Giunta delle elezioni del Senato, ha all'unanimità deciso che Nicola Di Girolamo siede illegittimamente in quest'Aula. Questo è il punto. E lo ha deciso con la forza di un rito che vede l'Aula poter intervenire sulla decisione della Giunta esclusivamente qualora venti senatori presentino un ordine del giorno per ribaltare quel deliberato. La decisione della Giunta ha, dunque, una forza che le viene non soltanto, appunto, dall'essere giudice esclusivo, ma ancora e di più dal Regolamento del Senato, che pone quella decisione come sovrana anche rispetto agli orientamenti dell'Aula e impone un comportamento - la presentazione dell'ordine del giorno - per tornare su quella decisione. Credo che dobbiamo partire da questo. Dobbiamo partire da questo e, probabilmente, commentarlo. Non lo farò con parole mie, Presidente: «l'intera vicenda dell'elezione al Senato di Nicola Di Girolamo costituisce un *vulnus* che colpisce la legalità e la costruzione istituzionale per la quale si è lottato quarant'anni in nome degli italiani residenti all'estero. La scelta di riservare loro il diritto di elettorato, sia attivo che passivo, è stata ampiamente valutata e condivisa e non può essere messa in discussione dalle posizioni strumentali non sono parole mie - di un mendace opportunista». La lettera è firmata dall'onorevole Mirko Tremaglia, al quale dobbiamo, come tutti sappiamo, l'iniziativa e la determinazione perché gli italiani eletti all'estero venissero rappresentati in questo Parlamento. E non vale la pena di tornare su una questione che pure ha sollevato il senatore De Gregorio. Non dobbiamo confondere i due piani: il piano della illegittimità del permanere il senatore Di Girolamo in Aula, da una parte, e l'altro piano, quello del riconoscimento al senatore Di Girolamo, non a Nicola Paolo Di Girolamo, della prerogativa dell'immunità nella sub-specie della negazione all'unanimità dell'autorizzazione all'arresto per i fatti che pure interferiscono con la sua elezione. Questa è la partita, Presidente. Una partita nella quale non possiamo trovarci a giocare più parti, ma dovremmo restare fedeli e stretti dal rigore con la quale la Costituzione ed il Regolamento descrivono e affermano i poteri del Senato. Noi siamo giudici e non possiamo essere gli avvocati del senatore Di Girolamo. A questo pensano prestigiosissimi avvocati di parte che, pure, su questo punto avevano deciso, come noi oggi proponiamo, che l'Assemblea E mi creda, Presidente: sento anche il peso di questa decisione per la ragione che, sulla base delle considerazioni che ci siamo scambiati in Conferenza dei Capigruppo, ciascuno di noi ha ripercorso all'indietro anche altre decisioni del Senato e della Camera dei deputati. Ciascuno, ovviamente, ricordava quelle che potevano essergli rimaste impresse per ragioni politiche in maniera più vivida. Io ricordavo i meno 11 deputati e il collegio imperfetto che per un'intera legislatura caratterizzò la Camera dei deputati o ricordavo una decisione piuttosto che un'altra; altri colleghi ne hanno giustamente e legittimamente ricordate altre, magari di segno opposto. Forse - lo dico con riguardo alla sua Presidenza e lei,

nel quale le istituzioni repubblicane vengono spesso fatte oggetto di dileggio e addirittura di disprezzo, anche da parte di molti cittadini e cittadine in cui il sentimento dell'antipolitica diventa ostilità nei confronti delle istituzioni e del loro procedere democratico,

avvertendo la responsabilità non soltanto nei confronti di noi stessi e dell'Aula, ma come ci tocca, visto che siamo rappresentanti del popolo italiano, anche del complesso delle istituzioni repubblicane e democratiche. Per usare un'espressione corsa anche tra noi, non credo che questa debba essere una occasione nella quale scorre il sangue. Probabilmente dovrebbe essere l'occasione nella quale recuperiamo vitalità, credibilità e affidabilità, nonché autorevolezza, al Senato della Repubblica.

Ciò, oltre che a sminuire l'importanza della Giunta, potrebbe costituire un precedente veramente grave per le istituzioni. Quindi, siamo contrari alla richiesta Signor Presidente, ribadisco la nostra richiesta di sospensiva, che nasce da una riflessione sofferta e responsabile che facciamo di fronte ad un caso inusuale. Non starò qui a ripercorrere i precedenti. In sede di Conferenza dei Capigruppo abbiamo avuto motivo di riflettere su tante decisioni che, sia al Senato che alla Camera, sono state prese su vicende

peraltro, a quanto mi risulta, non assunte all'unanimità (molti senatori hanno fatto richiamo a questa circostanza, ma diversi colleghi mi ricordano che così non è stato). Se ci fosse stata nel nostro Gruppo una valutazione divergente ci saremmo assunti la responsabilità di votare in quest'Aula anche in difformità dal parere della Giunta, cosa che non abbiamo fatto e non intendiamo fare e che la proposta di sospensiva non ci porta a fare. Dopodiché, non possiamo non ricordare

sulla composizione dell'Assemblea, ma avrebbe conseguenze di altra natura che il Senato giudicò eccessive lo scorso 24 settembre. Ecco perché abbiamo proposto una questione

Il rinvio alla Conferenza dei Capigruppo non corrisponde alla fissazione di un termine. Credo che la durata debba essere indicata in modo preciso. È soltanto su un termine preciso che noi possiamo essere chiamati a votare. Non possiamo essere chiamati a votare

la prego di tenere in considerazione queste nostre osservazioni.

ineccepibile la decisione della Presidenza di dare seguito a questa votazione accogliendo l'istanza del mio Capogruppo, avendo io confermato la relazione,

In mancanza di tali proposte, l'Assemblea non procede a votazione intendendosi senz'altro approvate le conclusioni della Giunta. Dichiaro aperta la

mi ero astenuto nelle considerazioni precedenti dall'affrontare i temi della relazione perché la discussione mi era parsa incentrata sulla questione dell'ammissibilità della proposta del collega Gasparri.

dai relatori Augello e Li Gotti. Colleghi senatori, per la prima volta nella storia d'Italia... parlo piano perché ho diritto alla stessa attenzione con la quale ho sempre ascoltato chiunque e mi sono sempre comportato in quest'Aula. Non volevo alzare la voce, perché questo è un argomento ampiamente riconosciuto e sottolineato dalla relazione dei senatori Augello e Li Gotti. Gliene do atto e li ringrazio, anche loro segnalano alla nostra attenzione che, per la prima volta nella storia d'Italia (non nella storia d'Italia repubblicana, ma nella storia d'Italia *tout viene all'attenzione del Parlamento una questione di ineleggibilità legata alla residenza. Dal 1865 al 2001 la residenza, con argomenti forti e motivati, è sempre e comunque stata ritenuta estranea alla nostra legislazione elettorale. È stata sistematicamente negata

e vi si è a suo modo adeguata l'opinione della Giunta. Devo dire però, onorevoli colleghi, che nella stessa relazione dei senatori Augello e Li Gotti,

non solo non vi siano indicazioni riguardo all'accertamento del requisito della residenza,

ritorno alla compostezza della mia citazione. Alla pagina 36 36 la relazione dice che nella legge n. 459 del 2001 non solo non ci sono indicazioni riguardo all'accertamento del requisito della residenza, ma viene del tutto ignorato il problema del contenzioso. Allora, con tutto il rispetto che non nego al presidente Follini, alla Giunta per le elezioni, ai relatori, alla maggioranza, all'unanimità e a come la Giunta, senza un passaggio in Aula, anzi con un passaggio in Aula del tipo di quello evocato questa mattina dal collega Gasparri, possa scegliere

Ho apprezzato, proprio perché non condividevo la sua relazione, che il collega Augello, con una dignità e una compostezza che lo onorano, in sede di questione sospensiva abbia detto

per la verifica dei poteri. Ecco, allora, che i profili di verifica dei poteri si sono sovrapposti ai profili di autorizzazione a procedere. Ho troppo rispetto di questa Aula, di ognuno di noi e del collega Di Girolamo e non voglio neanche evocare le implicazioni che l'accoglimento della relazione presentata dai senatori Li Gotti e Augello può produrre. A differenza di quanti ci richiamano alla sostanza a discapito della forma, io vi dico qualcosa che è di forma ma anche di sostanza. Il cosiddetto istituto dell'immunità (e, di conseguenza, dell'autorizzazione a procedere) non è né un privilegio, né una prerogativa, né un diritto del singolo parlamentare: è dell'Assemblea, per essere essa e soltanto essa arbitra (non giudice, me lo consenta il collega Sanna) della propria composizione. È stato in sede di verifica dei poteri che è iniziata una vicenda molto articolata, quella che dall'abate Sieyès ha portato il parlamentarismo medievale a farsi parlamentarismo moderno. Allora perché,

di interpretazione della norma costituzionale rispetto all'Aula? Ma che l'Assemblea

interesse di nessuno, ed era questo il senso della questione sospensiva, per la quale rimpiango non si sia registrato qualche consenso in più. Allora,onorevoli colleghi, rischiamo che la sovrapposizione delle prerogative del Parlamento in sede di autorizzazione a procedere sulle prerogative del Parlamento in sede di verifica dei poteri ci privi, quali che siano, delle virtù del subentrante Fantetti al resistente

parlamentare: una volta che ci sono un richiedente e un resistente, perché negare

«L'appartenenza ad un corpo politico elettivo come una Camera del Parlamento non può quindi essere pregiudicata dalla venuta meno del requisito della residenza

chi porta allora la Giunta a proporre all'Aula, con arrembante passo di giacobinismo, una conclusione nella quale si stabilisce che «La Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari

sollevata dal resistente, «propone al Senato (...) l'annullamento dell'elezione del senatore Nicola Paolo Di Girolamo»?

Presidente, colleghi, manifesto il mio imbarazzo per l'esito

che non rinnega il percorso procedimentale e decisionale con il quale si è giunti alla stessa, ma che oggi, tra altri colleghi, aveva sollecitato la Presidenza del Gruppo del Popolo della Libertà a richiedere la sospensiva su questo pronunciamento. Magari scendendo più nello specifico delle molte ragioni per le quali questa sospensiva era dovuta e necessaria, dovremmo ricordare ora, nel manifestare imbarazzo, che cosa rischia di accadere in seguito ad un voto erroneamente colorato di connotazioni politiche ed erroneamente presentato come una contrapposizione tra

Su questo medesimo fatto, che non rappresenta, nella sua valutazione e caratterizzazione giuridica, oggetto della competenza esclusiva della Giunta delle elezioni, il giudice ordinario è chiamato ad esprimersi. Il procedimento penale, che è in corso, dirà se Di Girolamo era residente o no in in quanto, se non lo era, a lui è da imputarsi il reato di falsa dichiarazione. La Giunta delle elezioni ha esaminato questo tema nello specifico, valutando un certificato di residenza, prodotto dal senatore Di Girolamo, proveniente dal consolato, che successivamente è stato revocato, ma che esisteva. Ha valutato l'esistenza di un contratto di affitto ed ha ritenuto, di fronte a fondate ragioni, che quel certificato di residenza non fosse valido e che il requisito soggettivo mancasse. Però, signor Presidente e colleghi, la valutazione sui requisiti di stato civile è rimessa alla giurisdizione esclusiva del giudice ordinario la Giunta delle elezioni oggi si trova ad avere definito, come conseguenza della propria decisione, la qualificazione giuridica di un fatto che un giudice domani potrebbe confutare. Nel nostro ordinamento non esiste la possibilità di revisione

che bisognasse attendere che il giudice ordinario, che ha competenza esclusiva, qualificasse il requisito della residenza. Non sfugge a nessuno che cosa capiterebbe in quest'Aula se domani venisse detto che quel certificato di residenza, rilasciato da un consolato e poi revocato, era comunque costitutivo del requisito necessario per la partecipazione alle elezioni nella circoscrizione Estero: Estero: avremmo fatto decadere un collega e non avremmo la possibilità di recuperare in revisione l'accertamento di un fatto che abbiamo assunto come presupposto nella Giunta delle elezioni, ma che non era di competenza della Giunta delle elezioni medesima. Dico questo, colleghi, perché la Giunta delle elezioni, nell'applicare in maniera correttamente analogica le procedure del diritto penale le procedure del diritto penale e del diritto civile, non ha potuto valutare tale questione, o forse distrattamente non ha potuto eccepire d'ufficio la valutazione che andava presentata una pregiudiziale in attesa che il giudice ordinario verificasse l'esistenza del requisito della residenza, perché il difensore di Di Girolamo, avvocato Taormina, in sede di decisione revocò la pregiudiziale,

colleghi - ed è la ragione per la quale il Senato ha sbagliato a non sospendere la decisione in attesa che il giudice ordinario si pronuncia su una materia di sua esclusiva competenza - che noi non abbiamo nessun meccanismo di revisione delle nostre decisioni. A noi non è consentito, neppure di fronte alla dimostrata insussistenza di un fatto che andava preso a presupposto di una decisione, di poter rivedere la decisione della decadenza. Qui davvero si crea un *vulnus* particolarmente grave, anche - e bene il Presidente del mio Gruppo a farlo presente - rispetto alla relazione tra questa votazione e quella che negò l'arresto. Chi lesse quella relazione - devo dare per scontato che tutti i colleghi l'abbiano letta - vedeva nella vedeva nella richiesta di arresto due elementi. Il primo: che esisteva un fondato motivo di commissione del reato di falso rispetto alla residenza. Il secondo: che Di Girolamo stava inquinando le prove perché stava producendo e ricercando la documentazione per far valere la propria residenza. Siccome questa seconda circostanza era palesemente vera, cioè era vero che Di Girolamo stava acquisendo i documenti per dimostrare la propria residenza, l'unica ragione per la quale il Senato non ha proceduto all'autorizzazione dell'arresto è perché nutriva dei dubbi sul fatto che la residenza non vi fosse. E questi dubbi erano fondati, perché al giorno dell'accettazione della candidatura, Di Girolamo aveva - giusto o sbagliato che fosse - un certificato proveniente dal consolato che attestava il fatto che era cittadino residente all'estero. Per queste ragioni esprimo particolare fastidio per il fatto che la discussione si sia

a coloro che nel mio Gruppo non hanno ritenuto di partecipare al voto, e di questo mi dispiace - entrare nel merito delle importanti, giuste ragioni che, per la dignità del Senato e per l'impossibilità di recuperare le nostre decisioni, stavano a fondamento della richiesta di sospensiva.

Grazie, signor Presidente,

alla fine, un voto per parti; anche se su questi argomenti ciascuno risponde esclusivamente alla propria coscienza, è abbastanza palese che la coscienza si è ripartita a secondo degli schieramenti.

convinti cioè che il senatore Di Girolamo avesse imbrogliato, avesse dichiarato ciò che non corrispondeva alla realtà e, in particolare, avesse dichiarato di possedere un requisito indispensabile alla candidatura e, di conseguenza, all'elezione nella circoscrizione Estero quando invece non ce l'aveva.

La relazione del Comitato inquirente, alla quale si è richiamato il senatore Augello

i quali mi è capitato di parlare è sostanzialmente sfuggito. I fatti sono questi. La norma della legge elettorale, sulla quale peraltro sono stati sollevati dubbi di costituzionalità

si debba essere residenti all'estero. Molti pensano che il trasferimento della residenza dall'Italia all'estero funzioni come un trasferimento di residenza da un Comune italiano ad un altro,

peraltro, giuridicamente dal momento in cui la richiesta è stata presentata - quel cittadino sarà effettivamente residente a Milano se prima era residente a Roma. All'estero non funziona allo stesso modo. Io sono stato iscritto all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero perché mi ero trasferito per un certo periodo all'estero; non ho mai avuto dal comune estero dove risiedevo

Il mio anno e mezzo di residenza all'estero è stato pertanto certificato unicamente da una mia dichiarazione presso il Comune nel quale risiedevo precedentemente in Italia e da nulla altro. Le norme sono state modificate in seguito, ma solo negli aspetti procedurali e non negli aspetti sostanziali. l'attuale senatore Nicola Di Girolamo, all'epoca evidentemente non ancora senatore, intendeva presentarsi all'estero, per avere evidentemente lavorato all'estero. D'altra parte, l'evidenza sta nel fatto che il senatore Di Girolamo ha preso 24.000 preferenze all'estero, segno, senatore Micheloni, che qualche presenza all'estero ce l'aveva e rappresenta l'estero esattamente quanto lei. *(Commenti del Mi meraviglio che lei, senatore, che fa parte dello schieramento che ha saputo esprimere grande sdegno per una battuta del Presidente del Consiglio sulla questione della violenza sessuale (che non aveva a mio parere nulla di offensivo)

Il senatore Nicola Di Girolamo, all'epoca, in tempi più che regolari, ha chiesto di trasferire la propria residenza in un certo indirizzo, che era assolutamente quello corretto, all'interno dell'area urbana di Bruxelles.

Coloro che vivevano nell'appartamento presso cui Nicola Di Girolamo ha chiesto di trasferirsi non sapevano che a quella via, a quel numero civico, non corrispondeva quel certo municipio, bensì quello accanto. In altre parole, l'appartamento è quello lì, la via è quella lì, ma, contrariamente a quanto coloro che hanno dato ospitalità a Nicola Di Girolamo

A questo punto, fatta questa domanda presso il Municipio sbagliato (ma riguardo l'unità abitativa, il luogo fisico giusto), il senatore Di Girolamo si è recato al consolato dicendo di aver fatto quello che esattamente aveva fatto, e cioè di avere preso residenza ad un certo indirizzo,

il mio indirizzo all'estero, senza che ci fosse stata alcuna certificazione da parte del Comune estero in cui io risiedevo, senza che ci fosse stata una certificazione e senza che io neppure sapessi esattamente dove si trovasse il consolato. - io fui regolarmente residente lì, al punto che il certificato elettorale mi giunse a quell'indirizzo. È allora corretta la procedura che si segue in quei casi, oppure è obbligatorio avere un'ulteriore prova? C'è un ulteriore argomento che sostiene che Nicola Di Girolamo, dopo aver fatto questa domanda e aver avviato la pratica presso il Municipio (purtroppo per lui, quello sbagliato)

questo ciò di cui stiamo parlando e, di conseguenza, non è la verità assoluta contro il falso assoluto. C'è chi ha dato un'interpretazione, secondo cui è indispensabile avere una documentazione completa ed essere registrati presso la municipalità straniera nella quale si intende prendere la residenza - nel qual caso

tutti noi sappiamo dov'è Bruxelles, ma credo che nessuno sappia dove si trova Etterbeek o Woluwe-Saint-Pierre. Credo che nessuno di noi lo sappia. Non lo sapeva esattamente neanche lui, pensava che il confine fosse un numero civico accanto.

il senatore Di Girolamo dalla sua carica di parlamentare, osservo che per questo gravissimo fatto - e cioè per aver segnalato il numero civico giusto, della via giusta e della casa giusta ma al municipio sbagliato - il senatore Di Girolamo non sarà più senatore e sarà soggetto all'arresto, questo Senato all'unanimità ha respinto pochi mesi fa. Questo è quello che stiamo giudicando. Io, membro della Giunta, ho partecipato alle votazioni. Ricordo che la votazione non ha avuto non ha avuto un esito unanime, contrariamente a quanto probabilmente nella fretta è stato ritenuto, ma questo è ciò di cui stiamo parlando. Questa è la responsabilità che ci si assume nel prendere questa decisione e direi che da questo episodio allo stupro e alla violenza del Parlamento c'è una bella differenza. Ricordo che qualche anno fa,

si decise con un voto a maggioranza che quello che aveva preso meno voti restava membro del Parlamento e che quello che ne aveva presi di più restava fuori dal Parlamento. Per la cronaca, il candidato che restò in Parlamento prendendo meno voti apparteneva alla sinistra, di cui è tuttora prestigioso esponente in quanto Presidente di una grande Regione. Vorrei pertanto invitare i colleghi ad

oppure non stabilire alcun requisito, visto che oggi chiunque risieda in Italia può candidarsi in una qualunque Regione, Provincia o Comune d'Italia.

grazie. grazie.

perché occorrerebbe liberarsi dai veleni che non da oggi circolano intorno a questa vicenda. vicenda. È a tutti noto che vi sono state una serie di iniziative pro o contro variamente qualificate, o squalificate, che hanno tentato di interferire con la decisione sovrana di questa Aula del Parlamento. Purtroppo, temo che anche a causa di tali pressioni in termini procedurali e di sostanza, che mal deporrebbe a favore di una accettazione *sic et simpliciter* della decisione della Giunta.

che la decisione dell'Aula è una decisione inappellabile, incensurabile, non soggetta a nessun gravame e che quindi quello che stabiliremo con il voto è qualcosa di definitivo. definito non riguarda i presupposti che dovrebbero giustificare un voto corrispondente a quello della Giunta, ma riguarda le conseguenze di un voto conforme a quello della Giunta, cioè l'estromissione definitiva di un parlamentare che, badate bene, non ha preso un voto meno di un altro e che è stato mal conteggiato. Ha preso, invece, più voti di un altro - tra l'altro appartenente al nostro stesso schieramento politico, per cui non facciamo questioni di interesse

tanto che la Giunta ha dovuto ripercorrere più strade prima di arrivare ad una decisione definitiva. Quali sono le due strade? Scontato che le questioni di eventuale eleggibilità riguardino la Giunta, si è prima percorsa la strada formalista, quella dell'esistenza dell'iscrizione all'AIRE, come prevede la legge attuativa del voto degli italiani all'estero, e non si è potuto negare che formalisticamente quella norma fosse stata salvaguardata. Se questi documenti sono stati formati in maniera illecita, non corrispondente al vero, ci sono altri soggetti, altre autorità, altre magistrature e non certamente la magistratura rappresentata in questo momento da noi senatori che possono eccepire, contestare o verificare questi dati. Formalmente la documentazione c'era e, ancorché revocata, nel momento in cui si sono presentate le liste elettorali e si è ammessa la lista al voto, non vi era nulla da discutere sul fatto formale della residenza anagrafica. Allora, la Giunta ha percorso l'altra strada, quella della residenza effettiva, agganciandosi alle norme del codice civile, in qualche modo contestando se stessa: se le leggi elettorali elettorali valorizzano il dato formale è chiaro che il dato sostanziale passa in secondo piano, come passa in secondo piano anche nel corso e nel corpo delle nostre elezioni nazionali. Guai se si aprisse per ogni questione di elettorato passivo o attivo una vicenda giudiziaria vertente sul fatto che l'elettore o il candidato risiedesse o meno in quel territorio, in quel Comune!

la Giunta non poteva e non può gestire queste vicende, come si possono gestire dinanzi ad un giudice civile, penale o amministrativo. questo sia un elemento fondamentale. rispettando naturalmente la sua decisione: quella della manifesta infondatezza della questione costituzionale. Presidente, riconosco le mie colpe e le mie responsabilità. Sono stato relatore al Senato sulla legge di attuazione e purtroppo, come molte leggi *bipartisan* - non tutte per fortuna - ma qualche volta...

È indubitabile che un problema costituzionale esista e posso testimoniare che si ritenne in quel momento prevalente, senza aver approfondito il dato costituzionale, il dato politico di un riconoscimento più forte ai cittadini residenti all'estero.

fonti di diritto pariordinate rispetto alla Carta costituzionale, e richiama leggi che hanno vigore in quei territori per dare attuazione a dei princìpi che comunque possono essere sostenuti da norme pariordinate alla Costituzione, in merito alle quali, fino a quel momento, non si sono mai sollevate questioni di costituzionalità. Ebbene, la Giunta ha svolto un giudizio preclusivo dichiarando, non la manifesta infondatezza ma l'assoluta fondatezza della costituzionalità del testo all'esame della Giunta stessa. essere tenuto presente, perché è evidente che per quanto riguarda l'elettorato passivo non esiste alcuna norma nei testi delle disposizioni costituzionali, introdotte nella Carta costituzionale con due separate decisioni del Parlamento, sulla quale possa poggiare il principio che l'elettorato passivo circoscrizioni estere possa essere negato a chi è cittadino italiano, come recita invece l'articolo 51 della nostra Carta costituzionale. E su questi punti devo dire che la valutazione della Giunta è lacunosa sotto tanti sotto tanti profili.

si sapeva che prima della scadenza naturale di quella legislatura non se ne sarebbe cavato un ragno dal buco. Questa è la realtà e lì si trattava di contare dei voti, non di stabilire se Tizio o Caio risiedesse o non risiedesse in quella

abbiamo deliberato di non concedere l'autorizzazione agli arresti del senatore Di Girolamo, e chiunque abbia letto ministero, autorizzata naturalmente dal GIP, ha ricavato una netta sensazione; anche se in questa Aula i toni sono stati dimessi,

forse per raggiungere qualche altro obiettivo. Credo che se l'Aula dovesse votare conformemente al parere della Giunta, ferma restando l'assoluta buona fede e trasparenza

nella procedura di riconoscimento dell'elezione del collega Di Girolamo. Questo è l'altro motivo per cui non voterò a favore della decisione assunta

Per quanto riguarda la questione pregiudiziale penale, va innanzitutto ricordato che davanti alla Giunta - e tutti abbiamo ritenuto molto correttamente - l'avvocato Taormina, difensore del senatore Di Girolamo, rinunciò alla pregiudiziale penale. infatti, ha sconfessato il presupposto di diritto su cui riposavano le indagini all'epoca in corso da parte della Giunta, in quanto quest'ultima non ha ascritto valore autocertificatorio alla dichiarazione resa dal Di Girolamo al consolato di Bruxelles il 14 febbraio 2008. La relazione della Giunta afferma che se che se l'eleggibilità riposasse sulla legittima iscrizione al registro AIRE non si potrebbe che concludere che il seggio del senatore Di Girolamo non è contestabile. In altri termini, il giudizio penale a carico del Di Girolamo non riveste alcuna influenza determinante sui risultati degli accertamenti della Giunta e non può trovare alcuna applicazione

di decadenza e in particolare di arresti domiciliari, che quest'Aula ha respinto circa quattro mesi fa, riguardava una serie di reati: false dichiarazioni al pubblico ufficiale, falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale, concorso in falsità ideologica, concorso in falsità in atti destinati ad operazioni elettorali, concorso in abuso di ufficio e soprattutto attentato contro i diritti politici del cittadino. Tutti questi reati, sui quali autonomamente procede l'autorità giudiziaria ordinaria, sono dipendenti dalla dichiarazione del 14 febbraio 2008 resa dal senatore Di Girolamo al consolato di Bruxelles. stessa dichiarazione invece non rientra assolutamente nella motivazione a supporto della proposta di decadenza dal seggio per il senatore Di Girolamo. Quindi, non è la dichiarazione al consolato belga a travolgere oggi il seggio del senatore Di Girolamo, ma è l'indagine svolta in maniera autonoma dalla Giunta in ordine alla residenza di fatto che - quale che fosse l'apparenza del diritto - come si è accertato mancava: Nicola Paolo Di Girolamo non era residente a Bruxelles il 10 marzo 2008, data di deposito delle candidature. L'articolo 8 della legge Tremaglia

che faccia saltare la partecipazione al concorso di un ordinario cittadino italiano. Quindi, prevedere una situazione di questo tipo per il senatore Di Girolamo ci pare quantomeno assolutamente fuori dalle norme costituzionali. Ripeto: l'accertamento della Giunta è totalmente indipendente dall'indagine penale e si poggia sulla base degli interrogatori che si sono svolti in Senato il 2 agosto e il 15 settembre 2008 davanti al Comitato inquirente, nonché su tutte le testimonianze che sono state acquisite dallo stesso. La proposta al nostro esame, che è stata votata a stragrande maggioranza - mi pare con un solo astenuto e un paio di senatori che si erano allontanati dall'Aula e non hanno partecipato al voto hanno partecipato al voto - deriva dall'affidabilità delle convincenti risultanze del Comitato inquirente e, pertanto, produce *ex se* l'effetto di annullamento dell'elezione in Senato di Di Girolamo. Per quanto riguarda i timori che sono stati espressi in quest'Aula, in particolare dal senatore Malan, in ordine ad un presunta ipotesi di arresto, innanzitutto segnalo che il Senato si è già pronunciato, con voti diversificati, contro gli arresti domiciliari che erano stati richiesti. Quell'indagine penale ha viaggiato autonomamente al di fuori di quest'Aula e da notizie giornalistiche pare ormai conclusa.

far decadere Di Girolamo dal seggio di senatore? È un problema di legalità. Bisogna rispettare la legge: tutti la devono rispettare, cominciando dai senatori fino ad arrivare a tutti i cittadini. Se non lo facciamo noi per primi, non possiamo pretendere che i cittadini rispettino la legge

il mio convincimento si basa su due argomenti di fondo. Il primo è un argomento relativo a quanto la Giunta mi ha fornito come elementi per poter valutare la relazione

Contemporaneamente, e sono costretto ad andare velocemente alle conclusioni per rispettare quanto il Presidente mi ha chiesto, mi sono dovuto anche interrogare, essendo un ingegnere, su un problema di sostanza e non di forma. Se avessi avuto un riscontro netto e nitido nella relazione della Giunta, io non sarei passato alla seconda fase; non avendo avuto questo convincimento netto e tenendo conto che sono in causa due persone con due interessi diversi, quello che mi sono dovuto chiedere è se vi fosse un discorso di sostanza. Il discorso di sostanza, per me, è quello relativo alla Costituzione, che dà ai cittadini il diritto-dovere di decidere dei propri rappresentanti. Nella stessa relazione sono messe in risalto le problematiche della legge Tremaglia, che quindi sono state prese in esame. La mia valutazione è che, tenendo conto di una relazione che non mi ha convinto,

senatore De Gregorio grazie.

Signor Presidente, il tentativo, sempre secondo le argomentazioni che illustravo qualche

che l'Aula si comporti in maniera garantista rispetto alla sorte del senatore Di Girolamo che, se fosse consegnato alla giustizia in questo momento, verrebbe rinchiuso agli arresti domiciliari. Mai le Aule del Parlamento, anche in caso di richieste di magistrati che hanno riguardato senatori e deputati dell'altro schieramento, si sono pronunciate a favore dell'arresto. Quest'Aula si è sostenendo implicitamente che i fatti non erano chiari, che bisognava approfondirli e cercare di capire quale fosse la responsabilità reale che il magistrato reale che il magistrato imputa al senatore Di Girolamo. Noi non smentiamo, con questo ordine del giorno firmato da più di 20 senatori e che richiama il nostro precedente appello, le decisioni della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari

affinché sia sospesa temporaneamente l'attività di verifica relativa all'elezione del senatore Di Girolamo fino a quando non sia stato conseguito un accertamento, con autorità di cosa giudicata, sui fatti oggetto del procedimento penale di cui citiamo il numero. Signor Presidente e onorevoli colleghi, la questione penale relativa al senatore Di Girolamo è assai delicata. Si Si tratta di fatti il cui accertamento in sede penale versa in una fase meramente investigativa, in cui il senatore Di Girolamo invoca la sicura non utilizzabilità delle risultanze investigative unilateralmente acquisite dal pubblico ministero, e conosciute dalla Giunta solo in ragione della loro considerazione per il diverso profilo della citata concessione dell'autorizzazione all'arresto.

che - lo ribadisco - possa non ribaltare le decisioni della Giunta, ma chiedere un maggiore approfondimento ai sensi di ciò che accadrà nelle aule di giustizia. avere il dovere di essere garantisti e che sia ingiusto consegnare all'arresto il senatore Di Girolamo. Chiediamo che questo approfondimento avvenga nella stessa sede della Giunta delle elezioni e delle immunità fino a quando tuttavia non sia stato conseguito un ulteriore accertamento. Mi appello alla coscienza dei colleghi, all'unità del Gruppo del PdL e ai garantisti dell'altra parte, che - lo so - sono tanti. Voglio ricordarvi, signori, che, qualche settimana fa, alla Camera abbiamo tutti insieme respinto, com'è accaduto in quest'Aula con il senatore Di Girolamo, l'arresto di un deputato del Partito Democratico abbiamo avuto la possibilità di sapere in breve che la scelta non era sbagliata, perché il tribunale del riesame ha respinto le ragioni per le quali il giudice chiedeva l'arresto. Voglio ricordarvi che queste Aule si sono comportate sempre e comunque in maniera ipergarantista. Non vorrei che la vicenda del senatore Di Girolamo dovesse segnare un precedente drammatico per le sorti di ciascuno di noi. Invito i senatori a respingere compatti questa possibilità, rinviando gli atti, quindi non smentendo nella sostanza le conclusioni della Giunta, ma aspettando un giudizio dell'autorità giudiziaria. Credo sia Credo sia una condivisibile aspirazione di tutti noi e chiedo all'Aula di esprimersi favorevolmente sull'ordine del giorno G1 da noi presentato. *(Applausi

Proverò a dire in pochi minuti perché, ad avviso del Gruppo del Partito Democratico, bisogna votare a favore delle conclusioni della Giunta e contro l'ordine del giorno De Gregorio. delle elezioni e delle immunità a quest'Aula sulla richiesta di arresto del collega Di Girolamo, qualche mese fa,

i requisiti che caratterizzano la tradizionale giurisprudenza, non solo di questo Parlamento, per l'applicazione di una misura restrittiva della libertà personale di un senatore. credo di avere le carte in regola per dirvi che, con eguale serenità, oggi possiamo ritenere verificati i fatti dimostrati nell'istruttoria della Giunta, acquisiti acquisiti mediante le testimonianze di testi liberi, davanti alle parti rappresentate dai loro assistenti legali, con l'assistenza tecnica con l'assistenza tecnica dei loro avvocati. Davanti alle conclusioni della Giunta, assunte con pressoché unanime e serena convergenza, noi, serenamente ripeto, possiamo ritenere valide

di mantenere nella sua titolarità il potere, enorme, tremendo che, ripeto, pochi Parlamenti al mondo oggi si attribuiscono, di valutare su se stesso, di giudicare i propri membri, di non attribuire ad un potere esterno la valutazione dei titoli di ammissione, cioè se uno di noi può stare o meno in quest'Aula. Possiamo anche rinunciarvi, colleghi, possiamo dire che questo compito, questo potere, questa prerogativa costituzionale non fa più parte del nostro tempo. Possiamo dire, però, che non siamo all'altezza di applicare l'articolo 66 della Costituzione?

volendo o non volendo non rileva, avesse il titolo per essere candidato nella circoscrizione Estero. Inoltre, il contenuto

nei contenuti della questione che ha preso il tempo del Senato fino a pochi minuti fa. Infatti l'ordine del giorno dice semplicemente, sconfessando completamente il lavoro della Giunta delle elezioni e che la Giunta doveva fermarsi nella valutazione del titolo di ammissione in questa Camera del senatore Di Girolamo una volta che aveva capito che su quei fatti era in corso un'indagine penale. Vi assicuro che questo noi l'abbiamo capito da subito, ma abbiamo anche affrontato il punto e abbiamo deciso che la questione penale, per quanto ci riguardava, non era determinante. L'abbiamo deciso proprio in ragione del fatto che, sul sul punto, abbiamo indirettamente dato ragione al senatore Di Girolamo dicendo che la dichiarazione consolare su cui si verte non è un'autocertificazione, quindi non aspettiamo un giudizio del TAR per dire se lui ha diritto o meno di rimanere qui

Il nostro esame si è limitato - ma è stato molto approfondito - a verificare se, in termini di sostanza, il senatore di Girolamo fosse o meno residente all'estero. I testimoni che hanno partecipato alla fase istruttoria, chiamati d'ufficio, alcuni chiamati anche a istanza di parte, non hanno confermato che il senatore risiedesse in quell'appartamento da lui stesso

spiacevoli, anche umanamente difficili da assumere, però qui, signori colleghi del Senato, la decisione da prendere è se siamo o meno all'altezza dell'articolo 66 della Costituzione. Vorrei concludere

che personalmente ritengo poco sopportabile, di sfrontatezza hanno argomentato in quest'Aula, senza il pudore di dire che avevano votato in un modo e che, si stava giudicando il loro lavoro, e sono diventati gli avvocati di una posizione che invece avevamo tutti insieme respinto in sede di giudizio. Essere all'altezza dell'articolo 66 della Costituzione significa anche mantenere alta

dell'esito finale di questo nostro voto daremo o l'abbrivio e una motivazione forte a quelle iniziative oppure manterremo nell'ambito delle nostre decisioni decisioni - umane, perfettibili, tutto quel che volete, ma assunte con il massimo della correttezza e della serenità e senza una motivazione di tipo politico - il potere e la prerogativa costituzionale di questo Senato. Lo voglio dire con parole che non sono mie, ma dell'onorevole Aldo Moro, che quando trattò questo tema nella Camera dei deputati ricordò ai suoi colleghi: «Una volta tanto non siamo legislatori, ma giudici, intendo giudici non in senso tecnico-giuridico, ma politico», ed è una scelta politica questa di mantenere in vita la prerogativa costituzionale di questo Senato. ancora: «Abbiamo dinanzi degli uomini e dobbiamo saper valutare con lo stesso scrupolo, con lo stesso distacco, con lo stesso rigore, i quali caratterizzano l'esercizio della giurisdizione. Perché anche noi, pur con tutti i nostri dibattiti politici, siamo oggi, se non nella forma, nella sostanza, dei giudici». Mi aspetto il giudizio sereno sul documento che la Giunta ha predisposto e vi ha proposto, colleghi, conseguenza del suo lavoro dei mesi scorsi.

però se vogliamo uscire fuori dall'ipocrisia, onorevoli colleghi, dobbiamo avere il coraggio di capire che qui non è soltanto un problema costituzionale; qui purtroppo, non certamente per responsabilità di quest'Assemblea, c'è qualcuno che, facendo una scelta, che forse il senatore Casson avrebbe fatto bene a ricordare, è entrato su una vicenda che si sarebbe potuta risolvere molto più serenamente senza inchiodare

Certo, avremmo potuto chiederci perché un magistrato abbia chiesto l'arresto di un senatore senza che questi - immagino - volesse scappare o, tanto meno, potesse occultare le prove o, peggio ancora, reiterare il reato. Però l'arresto Adesso è inutile che giriamo attorno ai dati costituzionali. Usciamo fuori dall'ipocrisia. Se qualcuno mi garantisce, ed è in condizione di farlo, che il senatore Di Girolamo con il mio voto non viene arrestato è un conto,

onorevole Presidente, per quel che mi riguarda non ci sarà un voto che possa condizionare l'arresto del senatore Di Girolamo. Un'utile mediazione potrebbe essere l'ordine del giorno G1, che rimanda ad una più giusta

il voto a scrutinio segreto per le votazioni riguardanti persone. Non vi è dubbio che nell'ordine del giorno che ci è stato sottoposto, sia nel dispositivo, dove fa riferimento esplicito Grazie,

ci illustra il significato del suo ordine del giorno spiegando che è volto ad evitare

Senatore Zanda, non vi erano da parte della Presidenza perplessità sull'ammissibilità del voto

anche questa volta sarò conciso. L'Italia dei Valori ritiene che l'ordine del giorno in

con queste parole: «propone al Senato - disattesa ogni diversa istanza - l'annullamento dell'elezione del senatore Nicola Paolo Di Girolamo». A prescindere della illeggibilità di alcune sottoscrizioni, magari qualcuna anche mancante, almeno nel testo che ho in mano fotocopiato - gli Uffici avranno - riteniamo impossibile un ritorno in Commissione per una verifica relativa all'elezione. La Giunta ha lavorato da mesi su questo punto, si è pronunciata e non mi risulta che nessun organo giurisdizionale,

così come mi pare, si debba introdurre surrettiziamente una sospensiva che l'Assemblea ha bocciato con un voto.

avessero concluso dicendo di votare contro la decadenza del senatore Di Girolamo, senza giri di parole più o meno contorti: la linearità questo imponeva e impone ad un'Assemblea che all'unanimità ha fatto una proposta tramite un organo quale è la Giunta, che ha concluso un percorso tecnico-giuridico, certamente con tutte le riflessioni di ordine politico che un organo del genere doveva fare. Per questo l'Italia dei Valori intende dare il proprio sostegno alla relazione ed alle conclusioni della Giunta ed esprimerà voto contrario sull'ordine del giorno G1.

Signor Presidente, colleghi senatori, abbiamo assistito a un dibattito nel quale si è sconfinato spesso e volentieri tra la forma e la sostanza. Abbiamo iniziato con un problema regolamentare; siamo passati, senza stabilire un confine, a parlare di problemi di sostanza; siamo tornati a problemi regolamentari, sentendo dire che nemmeno l'ordine del giorno (e non solo la sospensiva) sarebbe

Noi abbiamo cercato, in una situazione che è oggettivamente complessa e interroga le coscienze ma anche i convincimenti politici più profondi, di agire con equilibrio,

non abbiamo affidato un giudizio alla magistratura, ma abbiamo detto di voler acquisire ancora alcuni dati e alcune certezze. Soprattutto, dato premio a un formalismo astratto su un problema di sostanza. Non abbiamo dimenticato che quest'Aula ha votato contro l'arresto del senatore Di Girolamo su proposta della Giunta e a questo momento dell'*iter* giudiziario nessuno ci garantisce che il voto di oggi a favore delle conclusioni della Giunta non rappresenti una smentita di ciò che la stessa ci ha proposto. Noi non ci nascondiamo dietro un dito; sappiamo che dietro le pandette e gli articoli di legge ci sono degli uomini, e li abbiamo sempre considerati. Non vogliamo un'assoluzione; non vogliamo che si dica una parola definitiva su questa vicenda, ma vogliamo che tutti siano chiamati alla loro responsabilità. Non poniamo un problema politico di Gruppo: sappiamo perfettamente che in quest'ambito la coscienza ha un suo diritto e rimane libera. Ma ricordo che abbiamo sempre combattuto il formalismo giuridico per guardare alla sostanza dei problemi. É stata questa l'impostazione del nostro Gruppo sui problemi della giustizia che anche ieri, in questa Aula, abbiamo espresso. *(Applausi dal Gruppo* *PdL)*. Non intendiamo oggi smentire tutto ciò e abbiamo trovato una soluzione equilibrata per salvare

chi, secondo me in maniera poco elegante, ha ricordato Aldo Moro. Aldo Moro va ricordato fino in fondo; vanno ricordate anche le sue lettere dal carcere, che sono quelle che ci dicono

Signor Presidente, poiché dal testo che è stato diffuso non si evince la certezza delle venti firme, la pregherei di darci rassicurazioni in questo senso. PRESIDENTE. Sono tutti presenti.

Chiarisco all'Aula che, ove dovesse essere respinto l'ordine del giorno, si intenderanno approvate le conclusioni della Giunta nel senso dell'annullamento dell'elezione del senatore Di Girolamo.

Si vota sull'ordine del giorno del senatore De Gregorio che reca conclusioni difformi da quelle della Giunta. Lo ribadisco.

costituiscono opinioni espresse nell'esercizio delle funzioni parlamentari ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione. Chiedo al relatore, senatore Izzo, se intende intervenire. intervenire. Vi sono altri colleghi che hanno pari diritto al collega precedente che venga trattata la loro tematica, colleghi! Senatore Izzo,

Grazie, signor Presidente, e grazie anche per questo voto. Voglio ribadire che durante la conferenza stampa di cui si parla nel Documento non ho fatto alcun accostamento malizioso e non ho mai pensato né detto che il commissario dell'ente Fiera potesse essere il mandante delle telefonate che mi annunciavano l'imminente eliminazione fisica. Devo però dire che tutto quello che avevo denunciato attraverso un atto ispettivo firmato da me ma anche dal Capogruppo ha avuto riscontro nei fatti.

con ricorso del 24 dicembre 2003, il tribunale di Ancona - II Sezione civile ha sollevato conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato nei confronti del Senato della Repubblica in relazione alla deliberazione con la quale l'Assemblea, nella seduta del 26 novembre 2003, aveva dichiarato che il fatto oggetto del procedimento civile n. 659/01 R.G. pendente nei confronti di Augusto Cortelloni, senatore all'epoca dei fatti, riguarda opinioni espresse nell'esercizio delle funzioni parlamentari e in quanto tali insindacabili ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione. *(Doc. IV-quater, n. 18/XIV Leg.)*. Il ricorso è stato dichiarato ammissibile dalla Corte costituzionale con ordinanza 13 gennaio 2005, depositata in cancelleria il successivo 28 gennaio e notificata al Senato il 19 gennaio 2009. Nella seduta del 27 gennaio 2009 la Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari ha concluso all'unanimità nel senso che il Senato debba, per il tramite dell'Avvocatura dello Stato, costituirsi in giudizio dinanzi alla Corte costituzionale per resistere nel citato conflitto di attribuzione. Sulle conclusioni della Giunta può prendere la parola un senatore per Gruppo per dieci minuti. Poiché non risultano alla Presidenza richieste di intervento, metto ai voti le conclusioni della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari relative alla costituzione in giudizio del Senato della Repubblica dinanzi alla Corte costituzionale per resistere nel conflitto di attribuzione sollevato dal tribunale di Ancona - II Sezione

Tralascio un commento politico, perché non è questa la fase in cui esprimendo relativamente all'esito della vicenda, ma denuncio l'andamento sistolico e diastolico di attenzione rispetto alle nostre regole. Ebbene, il presidente Schifani che, per un caso della sorte, ogni volta presiede la seduta fino a quando non mi iscrivo a parlare sull'ordine dei lavori, aveva annunciato che entro martedì di questa settimana, cioè due giorni fa, avrebbe nominato d'ufficio due commissari, ancora mancanti per la costituzione della Commissione di vigilanza RAI. Oggi siamo a giovedì. All'università esiste il quarto d'ora accademico; le 48 ore senatoriali, visto e considerato che si va avanti di prassi in prassi e convenzione in convenzione, probabilmente si possono dare per acquisite. Ecco, sarebbe utile comprendere

precisamente mi riferisco, per comodità di consultazione degli Uffici, alla pagina 75 dello stampato. Al termine della interessante discussione sulle risoluzioni conclusive del dibattito

presente nella proposta di risoluzione n. 4. Laddove si parla delle circoscrizioni giudiziarie, al posto delle parole «sopprimendo i» i» (cioè sopprimendo i cosiddetti tribunali minori) vanno inserite le altre «con una razionalizzazione dei». Ora, siccome si tratta di una questione politica, ovviamente il senatore Casson, con pudicizia, l'ha smerciata come un refuso o un errore di battitura. Egli si è accorto del grande scivolone politico che, nei confronti di circa cento città italiane - dieci più, dieci meno - il suo Gruppo ha commesso, chiedendo la soppressione di importantissimi e nevralgici uffici giudiziari che fanno la qualità istituzionale della vita di queste città, ma lo ha fatto passare come un refuso.

Ah, siete dei pentiti?». Questa è la correzione, ma non fa niente, è tardi; sarò io a far conoscere a tutte le città italiane interessate che cosa dice il PD,

ma, poiché ritengo importanti, ai fini della polemica che andrò a trasferire su tutto il territorio nazionale e che è già in corso a carico del PD e dei suoi magistrati,

«Interviene il tale, gridando le tali parole») io chiedo che siano sbobinate dalla registrazione le mie testuali parole e siano inserite nel Resoconto stenografico.

il tentativo di assegnarci una volontà che non è quella che liberamente abbiamo manifestato. Non c'è possibilità di errore circa la nostra volontà: la nostra volontà è che si attivi un processo di razionalizzazione del sistema, il tema delle soppressioni è un argomento che non ci riguarda e che non ci appassiona. Piuttosto, su questo terreno, vedremo la maggioranza e il Governo cosa intenderanno fare e se i suoi disegni di legge e l'azione del Governo non mirino, invece, proprio all'operazione contraria, quella di anticipare, come viene fatto in alcune dichiarazioni, modalità di riorganizzazione che puntano alla soppressione; nel qual caso il collega dovrà battersi, e molto, all'interno di una maggioranza che, mi sembra di capire, ha più volontà di noi nella direzione delle soppressioni. Onorevoli colleghi, la Presidenza non può aprire in questa fase un dibattito di merito. Entrambi i senatori hanno puntualizzato e precisato; le loro puntualizzazioni saranno